L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994,

nella seduta pomeridiana del 19 marzo si è conclusa la discussione generale.

da un dibattito ricco e profondo, così come si è sviluppato all'interno della Commissione e come si è sviluppato la settimana scorsa all'interno di quest'Aula.

un testo che è entrato in 12a Commissione con equilibrio tra i vari disegni di legge che erano stati presentati, secondo una linea propria e definita della maggioranza. un testo basato sulla chiarezza nella formazione di alcuni princìpi (no all'eutanasia, no al suicidio assistito, no all'accanimento terapeutico) ha come conseguenza la non vincolatività delle dichiarazioni anticipate di trattamento e una chiarezza delle dichiarazioni espresse per iscritto, depositate e registrate. un testo che è stato migliorato grazie all'impegno di tutti quanti in Commissione e non solo, come ricordato dalla senatrice Bianchi, dall'impegno del Partito Democratico. In realtà, tutti abbiamo lavorato, maggioranza e opposizione; in particolare, è stata migliorata la parte riguardante il consenso informato, l'autodeterminazione, l'accanimento terapeutico. Ne è emerso senz'altro un testo più semplice, più chiaro; un testo che riduce significativamente i rischi di dubbi interpretativi. La settimana scorsa si è poi svolto in Aula un dibattito di alto profilo, del quale sento il dovere di ringraziare tutti, anche le persone lontane dall'impostazione del disegno di legge ma che hanno aiutato ciascuno di noi - e me in particolare - a riflettere, a trovare soluzioni migliori, anche attraverso una lettura più attenta degli emendamenti, o a volte a rinforzarsi nelle proprie convinzioni. L'ho affermato nella relazione la settimana scorsa e lo ha ribadito la senatrice Bonino in quest'Aula: il vero dibattito è sul significato della libertà, dei suoi limiti, della dignità della persona, sul significato del rapporto tra libertà e diritto. partendo dall'approfondimento di questi punti bisogna operare tutti quest'ultimo sforzo per giungere a una legge che sia la migliore possibile; una legge che possa raccogliere una condivisione più ampia possibile e che - come sollecitava il senatore Andria nel suo intervento - rappresenti il massimo equilibrio possibile; una legge che, fatti salvi i princìpi da cui parte, rappresenti una vera risposta laica e liberale, un punto d'incontro tra credenti e non credenti, basata sulla centralità e sulla dignità della persona.

Lo dice il disegno di legge, come anche la mozione n. 87 del 10 febbraio del Partito Democratico; lo dice l'emendamento principale presentato dal Partito Democratico su questo tema. Lo ripetiamo: idratazione e alimentazione non sono terapie, sono sostegno vitale e vanno garantite fino alla fine della vita. della vita. Vorrei ricordare anche in quest'occasione quanto detto dal senatore Lusi: «L'alimentazione e l'idratazione, anche artificialmente amministrate, devono quindi rientrare tra le cure normali dovute sempre all'ammalato, a patto che non risultino gravose per lui. Diversamente, la loro indebita sospensione può avere solo il significato di vera e propria eutanasia». Ancora, ci ricorda la senatrice Bianchi come la stessa Cassazione, definendo recentemente la nutrizione e idratazione artificiali come trattamento sanitario, ha dichiarato che «questo non costituisce oggettivamente una forma di accanimento terapeutico, ma rappresenta piuttosto un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale». ancora il senatore Lusi sottolinea come «considerazioni d'ordine generale permettono di credere che la vita umana continui fino a che le sue funzioni vitali - a differenza della semplice vita degli organi

Queste considerazioni - diceva il senatore Lusi - permettono di credere che la vita umana continui finché le sue funzioni vitali, a differenza della semplice vita degli organi, si manifestano spontaneamente o sia pure con l'aiuto di placente artificiali. Questo gran numero di casi forma oggetto di un dubbio insolubile ed essi devono essere trattati secondo quelle presunzioni di diritto e di fatto di cui abbiamo parlato.

cosa garantisce l'articolo 32 della Costituzione? Lo hanno ripetuto molti rappresentanti della maggioranza ed io lo voglio ribadire ancora una volta: garantisce la libertà di scelta delle cure.

Se scelgo di non farla sono certamente cosciente di accelerare un processo verso la morte; ma è un processo che lascia la storia naturale della patologia, che non interviene in maniera aggiuntiva sulla mia storia naturale. E se compio una scelta simile, ed ho la libertà di farla, il medico ha il dovere di rispettarla. Ma non si è liberi di eliminare quello che è sostegno vitale, quando questo non è terapia, che è cosa diversa da quando si cura una patologia. Né può diventare terapia per la sua forma di somministrazione. Non si è liberi di eliminare il sostegno vitale e richiedere poi una collaborazione al suicidio. Non si è liberi di scegliere se vivere o morire e, tanto meno, di chiederlo allo Stato. L'indisponibilità della vita umana risulta chiaramente dalle norme generali del nostro diritto, che puniscono l'omicidio del consenziente - articolo 579 del codice penale

E ancora, aggiungo, quale dimostrazione di volontà è forse più chiara di chi tenta il suicidio, di colui che decide di voler morire? E il nostro diritto certamente non condanna chi interviene, perché in quel caso non commette nessun reato di violenza privata, né alcuna violazione della libertà. Il senatore Marino e la senatrice Bonino sottolineano però che nel disegno di legge non è rispettata la volontà del paziente il senatore Veronesi aggiunge che il medico deve rispettarla, trattandosi di un principio deontologico. Ma dico di più: questo non solo è un principio deontologico, è un principio costituzionale che dobbiamo difendere, e lo abbiamo detto fino adesso. Attenzione

il presidente Nania; in quel caso il medico deve accettare e rispettare la volontà del paziente. Ma attenzione, il medico non eseguirà mai un intervento che non è necessario.

che in quel caso non vada rispettata la volontà del paziente e non possa essere chiesto al medico di fare ciò che deontologicamente e scientificamente è sbagliato.

per le persone e per la medicina e la scienza è cambiata. In quel caso il medico ha il dovere di riattualizzare quelle dichiarazioni e di dialogare con il fiduciario, cioè con colui che rappresenta la volontà, ma anche le ragioni e la ragionevolezza del paziente,

l'intervento è andato bene, ma vi sono state complicanze post-operatorie che si possono verificare anche con una certa frequenza; si è posta dunque la necessità di sottoporre il paziente ad una dialisi, anche temporanea, ma il paziente ha espresso nelle sue dichiarazioni la di non effettuare dialisi. Il chirurgo ne parla con il fiduciario, si rivolge poi al comitato etico e infine decide di rispettare la volontà del paziente.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono una fattispecie di atto medico, non sono come l'aborto che è una fattispecie in sé, per cui sulla base dei miei princìpi etici posso condividerlo o no e posso fare una scelta *a priori.* Sono realtà singole, per singole situazioni cliniche. Pertanto devo avere la possibilità di decidere caso per caso. Possono mai esistere obiettori di coscienza rispetto alle dichiarazioni anticipate di trattamento, come se fosse un fatto di principio? Io voglio rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento e non voglio andare oltre la volontà del paziente se condivido clinicamente quella realtà, se la scienza e la medicina non mi offrono nulla di diverso da quanto il paziente presumibilmente già conosceva. Altrimenti ho il dovere di dialogare con il fiduciario, di sforzarmi di parlargli, di offrirgli e prospettargli tutte le nuove soluzioni, se ritengo che queste possano essere utili, così come farei con un paziente cosciente e così come sono sicuro farebbe il senatore Veronesi con i suoi pazienti.

E arriviamo ad un altro punto cruciale: si è detto che questa legge vale per poche persone, quelle in stato vegetativo, ma vedo che vi sono alcuni emendamenti che ne propongono un ampliamento, La senatrice Bonino, però, si chiede cosa c'entrino i disabili gravi di cui ho parlato nella mia relazione: è proprio dei disabili gravi, senatrice Bonino, che stiamo parlando e mi meraviglio che, fino ad oggi, non ce ne siamo accorti; o forse si ritiene che una persona in stato vegetativo non sia più tale, ma solo un vegetale al quale non rivolgere più la nostra attenzione?

Voglio continuare a pensare - anche nel dubbio scientifico, che è ricerca e non certezza - che siano persone: persone con la loro vita, come diceva il senatore Lusi, e non solo vitalità biologica; persone con la loro dignità, con la loro dignità, disabili gravi, ed è intorno alla loro vita che dobbiamo legiferare con molta attenzione e con molta cautela. Senatrice Bonino, non penso di essere il solo a ritenere che la vita di un disabile grave abbia valore nella nostra esistenza: ho sentito e sento ancora il dovere e l'esigenza di richiamare quest'Aula, proprio ora, in queste ore, a questo tema, perché talvolta possiamo rischiare di dimenticarlo, nella speranza che tale richiamo possa aiutarci a riflettere e a prendere le giuste decisioni.

È vero che il nostro Paese è carente in questo settore, in particolare nell'Italia meridionale. È vero che la nostra popolazione va crescendo in età e l'accoglienza della disabilità deve essere uno dei temi principali di cui il nostro Governo si deve preoccupare. non continuiamo ad accusare la maggioranza di non aver voluto completare questa legge, perché è falso, e lo sappiamo tutti. La 12ª Commissione ha deciso all'unanimità la separazione dei due temi tra il Senato e la Camera:

che si continuasse a lavorare in parallelo e non vi fossero sfasature. So che la Camera sta lavorando, è a buon punto del suo lavoro e si è arrivati ad un testo base.

Sarà il completamento della nostra legge: solo così risponderemo a quel richiamo del senatore Gustavino, alle parole della canzone di Ligabue, ossia che non vorremmo mai scoprire che soli si viene e soli si va.

Signor Presidente, senatrici e senatori, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e hanno dato vita ad una discussione intensa, mai superficiale, di grande livello anche sul piano della civiltà dei toni. Il dibattito che si è svolto in questi giorni al Senato ha dato ragione a chi ritiene che nel Paese, come in Parlamento, il tema delicato della fine della vita sia stato approfondito e svolto in tutte le sue implicazioni e che debba ormai approdare ad una legge. Da circa dieci anni, infatti, si presentano e discutono disegni di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, mentre vicende come quelle di Piergiorgio Welby e, soprattutto, quella traumatica di Eluana Englaro hanno turbato l'opinione pubblica, sollecitandola a confrontarsi con il problema, al di là delle semplificazioni sullo staccare la spina, spingendo ciascuno di noi a informarsi, a distinguere e a maturare convinzioni meditate. Sulla necessità di dare un esito legislativo a questo lungo dibattito e di portare a compimento un *iter* parlamentare che più volte si è interrotto si sono espresse le massime autorità dello Stato, primo fra tutti il presidente Napolitano. Non farlo significherebbe alimentare i dubbi dei cittadini sulla capacità dei propri rappresentanti di svolgere con efficacia il compito legislativo rischiando di dare spazio a chi lamenta la tendenza del Parlamento a impantanarsi in discussioni senza sbocco, lasciando ad altri le decisioni. Fare una legge è più che opportuno: è necessario. Del resto è l'impegno che insieme abbiamo preso la sera in cui la drammatica notizia della morte di Eluana Englaro ci è piombata addosso mentre eravamo riuniti in questa stessa Aula. Oggi dobbiamo onorare quell'impegno, dimostrare che tra maggioranza e opposizione è possibile una dialettica accesa ma non paralizzante e che, senza per forza arrivare a posizioni comuni, si può però evitare di irrigidirsi pregiudizialmente in blocchi contrapposti. Il dialogo fra maggioranza e minoranza, infatti, c'è stato e può continuare. C'è stato grazie a chi da entrambe le parti ha voluto sfuggire al rischio del muro contro muro, non certo grazie a chi ha ceduto alla tentazione di atteggiamenti ostruzionistici. Le mozioni presentate la notte della morte di Eluana, per esempio, partivano entrambe dalla definizione di idratazione e alimentazione come sostegno vitale e non come terapie anche in Commissione, al di là di alcuni momenti di tensione, il confronto è stato utile: il disegno di legge è cambiato, come ha ricordato anche il relatore Calabrò, per esempio sul consenso informato, sulla durata delle DAT, sulla registrazione presso i medici di base. Ci può essere ancora spazio per ulteriori modifiche, sempre tenendo fermi i punti fondamentali su cui è costituita la legge e che voglio ancora una volta ricordare: la necessità di un consenso informato scritto e firmato, che non permetta di ricostruire a posteriori le volontà presunte di una persona non più in grado di esprimersi (come è accaduto per Eluana); un margine di autonomia per la valutazione del medico, che non può essere ridotto ad un ruolo di semplice esecutore o prestatore d'opera; la garanzia che idratazione e alimentazione non possano mai essere negate a nessuno. So che questo è un nodo fondamentale, anche se non mi è chiaro fino in fondo come una norma di garanzia sia diventata una frontiera, un terreno elettivo di scontro. Nessuno che sia in grado di intendere e volere vuole morire di sete. Non si tratta affatto di una dolce morte, come sappiamo tutti, ma di una agonia lenta e dolorosa. Perché dunque è diventato per alcuni l'emblema dell'autodeterminazione, l'espressione simbolica di una assoluta libertà personale? Più volte è stato fatto notare come i limiti a decidere sul proprio corpo siano ribaditi in vario modo nella nostra legislazione. Per esempio, nell'obbligo di indossare il casco, mettere la cintura di sicurezza o ancora nel divieto di vendere parti del proprio corpo o di automutilarsi. Tutti divieti incomprensibili e incongruenti se si dovesse partire davvero da una assoluta disponibilità di sé stessi. Se incontriamo qualcuno che vuole suicidarsi, cerchiamo di impedirglielo anche con la forza e sentiamo di aver fallito gravemente se non ci riusciamo. Eppure, un aspirante suicida ha certamente ragioni terribili e disperate per voler morire e queste ragioni il passante non può nemmeno conoscerle e valutarle: il gesto di impedire la morte è istintivo e pregiudiziale ed il fatto che chi sta per buttarsi da un ponte sia sicuramente autodeterminato non ci ferma. Temo che dietro il criterio dell'autodeterminazione agisca un altro criterio, non sempre esplicito e nemmeno sempre consapevole: quello della qualità della vita. Non si tratta tanto del dolore fisico, che ormai si può quasi sempre sconfiggere o enormemente attutire (voglio anch'io ricordare che presso la XII Commissione della Camera dei deputati è ormai in votazione un testo condiviso sulle terapie del dolore e sulle cure palliative): non si sceglie quasi mai la morte perché si soffre fisicamente in modo insopportabile. Piuttosto la si sceglie perché si ritiene la propria esistenza indegna di essere vissuta, la si ritiene una sorta di non vita. Il corpo che ti abbandona, si degrada, va per conto suo, è la naturale preparazione a quella cerimonia degli addii che tutti dobbiamo affrontare. Invecchiare e morire è sempre un percorso costellato da piccole e grandi incapacità, un progressivo scivolamento verso la non autosufficienza, verso la necessità di essere assistiti e aiutati come quando eravamo bambini. Se la vita e la sua qualità vengono identificate con l'integrità del corpo, con la piena autonomia, la delusione non può essere che immensa e inevitabile, perché siamo esseri umani che invecchiano, si ammalano, perdono l'autonomia fisica e mentale, e infine muoiono. Introdurre, magari in modo implicito, l'idea della qualità della vita è terribilmente rischioso; nello sforzo di cancellare il dolore e l'imperfezione, si può indebolire la solidarietà e la necessità della fratellanza umana. Il concetto di «qualità» applicato alla vita umana è pericoloso, non solo perché tende ad assimilare la vita a un bene di consumo, giudicandola secondo standard di tipo statistico, legati all'autonomia fisica e mentale, o alla capacità di svolgere alcune funzioni. Ma anche perché l'idea di qualità della vita nasce come espressione del giudizio soggettivo - sono io che giudico la mia qualità della vita ma finisce troppo spesso in una oggettività stabilita appunto da criteri medi, dalle leggi del mercato o da soggetti terzi. Quando si afferma di preferire la morte a una condizione di non perfetta capacità razionale, o a una condizione di dipendenza - e lo si è fatto anche in quest'Aula diventa più difficile affermare che ogni vita è degna di essere vissuta, che un grave disabile o un malato di mente possono condurre un'esistenza dignitosa come quella di una persona sana. Il male non si può cancellare, si può soltanto tentare di lenirlo, ripararlo, ed è questo il compito di chi sta vicino a una persona sofferente. Non c'è bisogno di credere in Dio per pensare questo, basta credere negli uomini. ci tengo a dirlo - è una legge di libertà, una normativa per applicare il tanto citato articolo 32 della Costituzione, che tra l'altro è quasi integralmente riportato nell'articolo 1 del testo Calabrò. Dobbiamo garantire la continuità dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, dunque la possibilità per il paziente di partecipare alla scelta della terapia anche quando non è più in grado di esprimere scelte, quando non sia cosciente e vigile, evitando il paternalismo medico e basandoci sul consenso informato. Si tratta di garantire la libertà di cura, stabilendo un confine che talvolta può essere sottile, ma deve sempre essere netto, con il «diritto a morire». Per questo è fondamentale stabilire cosa è terapia e cosa non lo è, e per questo idratazione e alimentazione hanno assunto un valore così fortemente simbolico. Tutti noi, in qualche momento della nostra esistenza, da piccoli, quando siamo malati o quando siamo per qualunque motivo incapaci di fare da soli, siamo affidati alla cura di chi ci vuole bene. L'accudimento, l'affidarsi nelle mani di altri è parte della nostra vita di relazione e nessuno può diventare adulto senza aiuto e cura. In inglese si parla di «*care*» e di «*therapy*», mentre in italiano il termine cura ha un doppio uso semantico e questo può generare confusioni: cura vuol dire terapia, ma anche accudimento. Distinguere, però, non è difficile: i gesti di cura non sono terapie, a prescindere da qualunque aiuto tecnologico. Non è terapia aiutare qualcuno nella mobilità, sia che gli forniamo la più tecnologica delle carrozzine, sia che semplicemente lo sosteniamo con le nostre braccia o lo accompagniamo. Non è terapia dare il latte a un bambino, anche se è latte artificiale, acquistato grazie a una ricetta medica, e somministrato con un *biberon*. Non è terapia qualunque gesto di accudimento, come vestire o coprire chi non può farlo da solo: eppure, se non lo facciamo, una persona può morire di freddo. Esiste, in questo senso, la più semplice delle controprove su cosa sia o non sia terapia: se un malato di una qualunque patologia, per esempio un tumore, sospende la propria terapia, morirà di tumore; se lo stesso malato sospende idratazione e alimentazione, magari fornita col sondino, non morirà di tumore, ma di disidratazione e denutrizione. Questa differenza vale anche per la ventilazione, di cui si è chiesto più volte in quest'Aula. Voglio ricordare che su questo punto, cioè se idratazione e alimentazione siano o no terapie, non c'è accordo nella comunità scientifica, contrariamente a quanto alcuni hanno detto. Talvolta, chi chiama più decisamente in causa la scienza, trascura di accertare se la scienza sia concorde, oppure trascura di ricordare le ultime acquisizioni scientifiche. Penso a quante volte ho sentito parlare di «stati vegetativi permanenti» o di «irreversibilità», definizioni che da tempo non sono più adottate per le persone in stato vegetativo. Sappiamo pochissimo, in realtà, dei malati ritenuti in condizione di incoscienza, tanto che recenti ricerche hanno dimostrato un'insospettata attività cerebrale in alcuni pazienti in stato vegetativo: sono persone che "sentono", che trattengono, in qualche remoto angolo della mente, emozioni, immagini e ricordi. Tutti quelli che hanno avuto una persona cara in coma o in stato vegetativo conoscono bene l'ansia con cui si spia un segno, si cercano le tracce di un riconoscimento, un guizzo di coscienza; e se quel segno tanto atteso non arriva, nessuno può davvero assicurare che ogni rapporto sia reciso e che una carezza, una voce non suscitino una risposta silenziosa. È grave non riconoscere in questa condizione una forma di disabilità estrema, come sostengono del resto tutte le associazioni dei familiari di persone in stato vegetativo. È grave parlare di «mera vita biologica», senza adottare nemmeno, come ha ricordato il ministro Sacconi, il laicissimo principio di precauzione. Non è l'incoscienza, anche duratura, a non rendermi persona. Lo Stato vegetativo non coincide con la fase terminale delle vita ma solo con una patologia estremamente invalidante, qualcosa verso cui dovremmo avere un di più e non un di meno di cautela e di rispetto. Il limite su cui tutti possiamo concordare è quello dell'accanimento terapeutico che, però, acquista significato solo quando una persona è avviata verso la morte naturale. Ed è questo il senso anche della lettera erroneamente attribuita a Paolo VI, che ho sentito mille volte citare negli ultimi giorni. Autore e firmatario della lettera è, in realtà, il cardinale Villot e non il Pontefice. Ma il senso era proprio nel deciso rifiuto delle terapie sproporzionate nel momento in cui ci si avvia verso la fine della vita. Un limite ragionevole e condivisibile, con cui concorda il sentimento di fratellanza che tutti condividiamo e che ci fa riconoscere nella morte non un momento di libertà ma il cuore della condizione umana e della sua intrinseca fragilità e limitatezza.

le relazioni, più ci penso e più mi convinco che faremmo cosa utile e saggia se ci prendessimo un periodo di riflessione, perché credo - lo abbiamo sostenuto già la settimana scorsa - che in realtà questa legge contraddittoria e pasticciona non solo è incostituzionale, ma stabilisce una sorta non di diritto alla vita, bensì di obbligo di vivere obbligo di vivere e una sorta di scienza di Stato. Che vogliate o non vogliate considerare l'alimentazione e l'idratazione forzata terapia o meno, voi stabilite che devono essere obbligatorie per tutti, in qualunque condizione, e che quindi non vi è libertà di esercizio che possa essere data al cittadino. Non la farò lunga per via dei tempi. Però, vi prego di riflettere ancora un momento. Questa legge cambia nella sostanza il rapporto individuo-istituzioni - ripeto - questa legge cambia e cambierà d'ora in poi il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Penso che a molti venga il dubbio che quando lo Stato entra nel letto degli sposi, degli amanti o dei malati non è un gran bel giorno, in particolare se questo vuol dire che chi ci sta non è più libero di scegliere. Allora, signori colleghi, fino all'ultimo mi adopererò affinché questa legge non possa vedere la luce. l'idea di molti è che intanto si salva la faccia al Senato e poi, nel passaggio tra le due Camere, si vedrà di ripensarci meglio. Penso che sarebbe bene non arrivare neanche alla votazione al Senato e prenderci tutti una pausa di riflessione non sugli aspetti sanitari, ma su quelli che attengono all'individuo e alle sue prerogative. Per questo,

Non è uno strumento messo in mano al medico: è lo Stato che organizza le regole per poter rispettare al meglio l'inviolabilità e l'indisponibilità della vita. Per questo chiediamo all'Aula di procedere

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, in riferimento agii articoli da 01 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 01.4, 01.6, 01.20, 01.36, 01.38, 1.221, 1.274, 1.277, 1.278, 4.67, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 8.0.2, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.70 e 4.77. Resta sospeso il parere sull'emendamento 1.269 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 9». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia soppresso l'articolo 5».

colleghi, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili per estraneità all'oggetto della discussione gli emendamenti concernenti la sperimentazione scientifica (01.1, 01.2 e 01.3) e la disciplina della cure palliative (01.20, 01.261, 5.0.1 e 5.0.3). Sono inoltre improponibili l'emendamento 7.120, in quanto non formulato in termini generali ed astratti, Sono inoltre improponibili l'emendamento 7.120, in quanto non formulato in termini generali ed astratti, l'emendamento 7.104, contenente un riferimento a un Capo di Stato estero, nonché gli emendamenti 1.68 e 1.91 in quanto privi di contenuto normativo. prima di passare all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, avverto che da parte del prescritto numero di senatori sono pervenute diverse richieste di votazione a scrutinio segreto su articoli ed emendamenti al disegno di legge al nostro esame. La Presidenza ha valutato tali richieste secondo i criteri che seguono. L'articolo 113, comma 2, del Regolamento stabilisce che «l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano». Ogni altra forma di votazione costituisce dunque una deroga rispetto a quella ordinaria e ha carattere residuale. Le disposizioni relative devono essere considerate in questa prospettiva e sono perciò di stretta interpretazione. Per quanto in particolare concerne lo scrutinio segreto, ricordo che - come appare dai lavori preparatori - la modifica regolamentare del 1988, che condusse al testo attuale dell'articolo 113, fu dettata proprio dall'intento di circoscrivere a casi rigorosamente determinati l'area delle votazioni segrete. Sia dalla lettera del Regolamento (carattere normale della votazione per alzata di mano) che dalla storia e dalla *ratio* delle norme sullo scrutinio segreto si ricava che esso può essere ammesso non per tutte le deliberazioni che implichino genericamente i diritti di libertà relativi ai rapporti civili ed etico-sociali previsti dagli articoli della Costituzione richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Regolamento, ma solo per quelle che abbiano per effetto la limitazione o la compressione dei diritti stessi. In questa occasione, peraltro, la Presidenza ha fatto un'applicazione di questi criteri flessibile e rispettosa dell'esigenza dì consentire una compiuta e libera espressione del voto su argomenti di particolare delicatezza, che toccano tanto da vicino la coscienza individuale. Pertanto comunico che, per il disegno di legge in discussione, lo scrutinio segreto è stato ammesso per circa la metà delle richieste formulate e in particolare con riguardo a: l'autodeterminazione rispetto a condizionamenti politico-religiosi, il dissenso su atti medici, il rifiuto delle cure e dei trattamenti sanitari, la revoca del consenso ai trattamenti sanitari, l'eutanasia, l'accanimento terapeutico, la tutela dell'infanzia, il consenso dell'incapace, il carattere vincolante della dichiarazione anticipata di volontà, l'idratazione e la nutrizione, l'obiezione di coscienza del medico, il contrasto tra medico e fiduciario, le fattispecie in cui venga disattesa la volontà del paziente, le modifiche al codice penale. L'elenco degli emendamenti e degli articoli ammessi al voto segreto, come pure di quelli non ammessi, entrambi con le relative motivazioni, è già stato distribuito ai Gruppi ed è a disposizione degli onorevoli senatori. Per quanto riguarda la richiesta di scrutinio segreto sulla votazione finale del provvedimento, la Presidenza si riserva di valutarla all'esito dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G101, si propone la seguente riformulazione:

trattamento, impegna il Governo a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più schemi di provvedimento, da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le seguenti finalità:

Signor Presidente, senatrici e senatori, signori membri del Governo, il Gruppo del Partito Democratico ha deciso di sostenere l'ordine del giorno G100, che vede come perché, con senso di responsabilità verso i cittadini italiani, siamo convinti che le cure palliative debbano essere garantite a tutti. Oggi non è così e infatti, dei 98 *hospice* presenti sul nostro Paese, 87 operano nelle Regioni del Centro-Nord e solo 11 in quelle del Sud. Per fare un esempio, signor Presidente, 38 si trovano in Lombardia e soltanto 3 in Sicilia. In una società come la nostra, in cui la morte avviene nella gran parte dei casi al termine di una lunga e debilitante malattia, poter contare su strutture specializzate nell'assistenza nelle fasi terminali è di grande sollievo per i malati e per i loro familiari. E per la nostra sanità pubblica, costruita sui princìpi di equità e di solidarietà, offrire questo tipo di servizi dovrebbe essere un dovere! È importante ricordare a tutti che in Italia non vi è una formazione specifica dei medici rispetto alla complessità delle cure palliative, dato che non si apprendono all'università, e anche questo fa sì che tutto il sistema abbia urgente bisogno di un intervento da parte del legislatore. Tuttavia, gli emendamenti presentati su questa importante materia in Commissione sanità sono stati dichiarati inammissibili e noi crediamo che questo sia un fatto grave, che testimonia il totale disinteresse della maggioranza verso i problemi dei più deboli e dei più bisognosi. La maggioranza ha fatto riferimento ad un accordo informale con la Camera dei deputati che sta lavorando su un disegno di legge relativo alle cure palliative. Sinceramente, vorrei chiedere ai senatori del centrodestra se i cittadini italiani, per cui tutti noi lavoriamo, possano capire che un accordo informale tra i due rami del Parlamento è più importante di una risposta concreta ai loro problemi oggi, non domani. Ci auguriamo almeno che quel disegno di legge sia condiviso, non come la legge che stiamo votando questa settimana e, soprattutto, che segua un *iter* altrettanto rapido di quello seguito al Senato per approvare la legge sulle dichiarazioni anticipate di volontà. Personalmente non sono molto fiducioso che andrà così. Temo piuttosto che il capitolo degli *hospice*, delle cure palliative e delle terapie del dolore sarà ancora una volta rimandato o, meglio, demandato alla capacità delle singole Regioni di rispondere in maniera autonoma alle esigenze dei cittadini di quel territorio. Mi auguro sinceramente di sbagliarmi e che questo importante ordine del giorno rappresenti davvero un impegno e un'assunzione di responsabilità precisa per il Governo.

e diventano estremamente poco liberi in rapporto all'altro mondo che è loro davanti. Credo che in Italia si debba fare molto, come diceva prima il senatore professor Marino, non dimenticando che i primi *hospice* furono deliberati nel 1998.

non solo malati terminali, che necessitano di un sostegno economico per poter accedere a questo genere di cure particolari, ma anche quei malati gravi che presentano malattie rare, che non trovano integrale tutela da parte del Servizio sanitario nazionale e che alimentano quella cultura dell'abbandono che con questo ordine del giorno e questo disegno di legge intendiamo contrastare.

alcune questioni. Il disegno di legge su cui ci siamo esercitati propone sicuramente l'idratazione e la nutrizione come sostegno vitale e come accompagnamento garantito a questi pazienti fino alla fine della vita. È chiaro che il provvedimento si rivolge soprattutto ai pazienti in coma, per quanto riguarda il sostegno vitale, e ai pazienti in stato vegetativo più che al malato terminale, di cui ci si è occupati nel precedente ordine del giorno.

doveva prendersi carico anche di questo aspetto, cioè della cura del paziente sul territorio e nelle famiglie, del paziente reale che soffre insieme alla sua famiglia. Questo non è successo e con questo ordine del giorno vogliamo almeno impegnare il Governo perché se ne faccia carico e perché venga istituita una rete vera e propria per la cura e l'assistenza di questi pazienti, una rete che dia a tutte le Regioni un percorso garantito e uguale, così come vengono garantite idratazione e nutrizione. Noi dobbiamo assolutamente far sì che questi pazienti siano presi in carico dal sistema sanitario pubblico e che le nostre famiglie italiane siano aiutate in questo difficile percorso di sofferenza.

tantissimi sono i malati che hanno bisogno di questi ausili tecnologici per garantirsi una qualità della vita accettabile. Vorrei ricordare che nella passata legislatura l'allora ministro Turco stanziò 10 milioni di euro per questi dispositivi e che tali fondi sono stati bloccati, come tra l'altro ricorda anche la senatrice Boldi nell'ordine del giorno Questo, naturalmente, ha causato una diversa distribuzione ed erogazione nelle varie Regioni italiane. Soltanto tre Regioni hanno stanziato, ad oggi, risorse per tali dispositivi.

infatti, di una situazione nella quale, una volta tanto, i fondi ci sono, perché sono stati stanziati e finalizzati,

perché ci facessimo portatori di questa istanza, chiederei di fare al più presto tale ricognizione per cercare di capire per quali ragioni moltissime Regioni non hanno ancora iniziato la distribuzione dei puntatori oculari.

tale perdita di dignità della vita da ritenere che sia meglio non vivere la vita che stanno vivendo e chiedere addirittura di

la cura dello stato vegetativo come livello essenziale di assistenza. A me sembra importante stabilire in questo disegno di legge il diritto delle persone affette da queste patologie; anche se qualcuno ha posto degli ostacoli di ordine contabile, credo che

Signor Presidente, non vorrei che si innescasse un meccanismo di marchio d'infamia per cui i documenti sottoscritti dai radicali vengano scansati a prescindere. L'ordine del giorno G103 affronta una questione fondamentale relativamente ai costi di gestione che la pubblica amministrazione si assume si assume tutte le volte che vengono utilizzati dei programmi *software* proprietari. Chiediamo di poter utilizzare il *software* libero, che non ha necessità di pagamento di licenze, per la creazione del Registro nazionale delle dichiarazioni inoltre che ci si avvalga della collaborazione partecipativa e gratuita degli sviluppatori di questo tipo di programma e di utilizzare in maniera multimediale quanto più possibile la pubblicizzazione dell'esistenza dello stesso. Il ministro Brunetta proprio l'altro ieri ci ha invitato a spengere le luci e i computer quando abbandoniamo le Aule. Sicuramente vi sarà un grande risparmio relativamente al consumo di energia elettrica, ma se iniziassimo ad utilizzare

è a carico del Sistema sanitario nazionale, l'altro 50 per cento è a carico degli enti locali, che possono rivalersi sull'assistito in base al suo reddito. Purtroppo, a causa della mancata adozione di un decreto ministeriale, atteso dal 1998, i Comuni e gli enti locali si comportano in maniera disomogenea: alcuni si rivalgono sull'assistito, altri sui familiari.

Sono oltre 120 - ripeto - i cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa. Alcuni dei loro emendamenti sono stati presentati così come li abbiamo ricevuti, altri hanno necessitato di un lavoro di affinamento. Questo è il primo ringraziamento. Le nostre proposte premissive, presentate in numero superiore agli emendamenti che abbiamo presentato all'articolato, vogliono in qualche modo riassumere quello che, secondo la delegazione radicale nel Gruppo del PD, dovrebbe essere al centro di un testo che ha l'ambizione di voler diventare un testamento biologico: in che si riconoscano come vincolanti le volontà e non gli orientamenti del paziente; che si risponda, quindi, agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione italiana, cioè che si adotti un testo che obbedisca alla nostra Carta, ma soprattutto che si codifichi un testo che non sia antiscientifico, per cui il sostegno vitale - questa nuova formula che è stata utilizzata per mantenere in vita perennemente anche chi è in fase di malattia irreversibile - venga trattato come tale, cioè come una formulazione antiscientifica, e che si includa nella possibilità di espressione della volontà anche quanto riconosce l'articolo 32 della nostra Costituzione, cioè la possibilità di sospendere i trattamenti. Questo vale per il merito degli emendamenti. Per quanto riguarda, invece, il merito del dibattito politico,

nel congresso di Alleanza Nazionale, tenutosi lo scorso fine settimana, è parso finalmente di capire che esiste un altro tipo di interpretazione del termine libertà che voi della maggioranza avete voluto mettere nel nome del vostro partito. Mi riferisco, in particolare, a quanto affermato dal presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha centrato tutto il suo intervento sull'individuo, sull'autodeterminazione e sul fatto che la libertà individuale venga prima del cosiddetto bene pubblico. Ebbene, dispiace sapere che i senatori del Gruppo PdL non praticheranno la loro affermazione di coscienza perché è stato suggerito loro di ricordare che, in futuro, potrebbero avere problemi ad essere inclusi in lista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

non può essere nutrita forzatamente, ma si deve avere il suo consenso; questo vale per la persona capace. Vi chiedo di votare almeno questo emendamento, poi proporrete nella legge che la persona incapace di intendere e di volere debba invece essere sottoposta ad

assistito. Bene, vogliamo invece incominciare ad affrontare l'argomento dell'eutanasia nell'unico modo in cui un Parlamento dovrebbe fare, cioè normandolo, disciplinandolo, legalizzandolo e, appunto, legiferando, in maniera da poter porre limiti e norme, perché il paziente veda rispettata la propria volontà.

1**, inserire il seguente: «Art. 01. 1. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana, nel rispetto della volontà dell'individuo.

la possibilità di costruire un periodo con soggetto e predicato e la seconda che resta preclusa con una sorta di *capitis deminutio*.

vorrei capire bene cosa stiamo votando, perché a mio avviso vi sono state una decina di votazioni in cui ciò che è accaduto non è rispondente neanche alla logica della sintassi prima che a quelle della politica.

e l'idratazione fornite in certe condizioni e a certi soggetti sono trattamenti medici. Lo abbiamo già detto prima. Il codice deontologico riconosce la facoltà del paziente di non essere sottoposto ad alimentazione ed idratazione contro la sua volontà. L'appello è che anche quest'Aula riconosca quella che è la realtà. Poi, se vogliamo dire che questa non è carta

in altro momento chiederò una convocazione della Giunta per il Regolamento su questo punto. Colleghi, intervengo perché credo che sia

politiche, personali e culturali dalle quali provengono. Sono emendamenti che nascono da una discussione molto lunga fra noi e anche da una capacità di mediazione che non vorrei sembrasse di rito e che vorremmo offrire alla discussione dell'Aula e anche dei colleghi C'è poi una serie di emendamenti che nasce dalla piena libertà di coscienza di alcuni dei nostri colleghi ed alcuni di questi sono sottoscritti da un numero consistente di senatori.

Voglio spendere pochi secondi per spiegare una cosa ai colleghi della maggioranza, anche perché lo devo a quanti hanno lavorato all'ipotesi di quelli che noi chiamiamo emendamenti condivisi, cioè riconducibili all'intero Gruppo parlamentare.

e di sfuggire ad un senso comune, che pure dovrebbe esserci quando si usano parole che appartengono al patto sociale che è la Carta costituzionale. Le faccio un esempio, sottosegretario Roccella:

di mostrare anche le nostre differenze, perché sapevamo che c'erano e che non avevamo alibi né scorciatoie. E non abbiamo avuto bisogno di scrivere nessuna lettera per coniugare, o meglio piegare, la libertà di coscienza Gruppi PD e IdV).* Noi siamo qui per quello che siamo: uomini e donne liberi, che hanno svolto un lavoro difficilissimo e che oggi presentano la posizione del Gruppo del Partito Democratico. Uomini e donne liberi, che celebrano la libertà di ciascuno su questi temi

complesso e importante che riguarda tematiche certo non ordinarie e che, quindi, chiama in campo non solo i Gruppi parlamentari, come articolazioni del dibattito democratico ma, mai come in questo caso, la coscienza dei singoli. Finocchiaro, visto che ha citato una lettera, che ha fatto bene il Presidente del Consiglio ad assumersi la responsabilità di una valutazione che il Governo aveva già fatto emanando un decreto. Non voglio riaprire discussioni che sono consegnate alla storia del dibattito parlamentare e costituzionale. Nella lettera si

Il nostro Gruppo, però, ha un orientamento, ha sostenuto l'azione del relatore, del Presidente della Commissione e di tanti colleghi. Quindi, rispettiamo la libertà di ciascuno, ma siamo orgogliosi del lavoro svolto e del fatto che sia condiviso anche da chi guida una formazione politica e il Governo della Repubblica italiana. Presidente, colleghi, il Gruppo ha lavorato con grande passione ad una legge che gli italiani vorrebbero la migliore possibile. Abbiamo cercato ogni forma di utile mediazione, superando gli ideologismi che hanno pervaso la discussione anche in Commissione.

non solo la nostra parte politica, ma tutta l'Assemblea, che ha interesse a fare la migliore legge possibile e non una legge quale che essa sia. Per questo continueremo con pervicacia e con passione a collaborare in quest'Aula per migliorare un testo che al momento non ci convince.

mio avviso, partono sempre da equivoci che è nostro compito chiarire. Nella legge si fa riferimento, in via di principio, alla circostanza - dal mio punto di vista molto importante - che si dà attuazione agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Con gli emendamenti da me presentati chiedo che sia meglio specificato quando si fa riferimento ad una norma in attuazione dell'articolo 2, quando si fa riferimento ad una norma in attuazione dell'articolo 2, quando invece si fa riferimento ad una norma in attuazione dell'articolo 13

alla tutela del diritto alla vita, e il riferimento all'articolo 32, che riguarda la tutela della salute e che, come stabilisce in maniera chiara l'Organizzazione mondiale della sanità, non va inteso come diritto a vivere, ma diritto a vivere bene. Si può anche ritenere che la nostra Costituzione sia inattuale, soprattutto nei princìpi generali. D'altronde, indirettamente la presidente Finocchiaro

tra diritti inviolabili dell'uomo da parte degli altri e diritti inviolabili da parte del suo titolare. Si può anche sostenere che i Padri costituenti non

piuttosto del fatto che il diritto alla vita è inviolabile da parte degli altri e da parte del titolare della vita. Pertanto, ci si deve adeguare a questa circostanza. Ecco perché, concludendo il mio intervento sugli emendamenti, vorrei ribadire con forza che una cosa sono i trattamenti sanitari che attengono al diritto alla salute, cioè al diritto a vivere bene, altra cosa sono tutti gli atti che attengono al diritto inviolabile alla vita. Ribadisco con forza anche che bisogna adeguarsi con la legge alla Costituzione

salvo che la legge non disponga altrimenti. Proponete questa modifica, discutiamone, ma in ogni caso nella Costituzione questa modifica non è e quindi io dissento (tra virgolette) da questa maggioranza di centrodestra che si è dimostrata molto "aperturista" nei confronti di richieste del centrosinistra che non sono né previste, né tollerate dalla nostra Costituzione

venivano da una scuola che conosceva perfettamente il diritto e quando hanno definito il diritto alla salute fondamentale e il diritto alla vita inviolabile sapevano esattamente quello che dicevano.

dal giorno famoso della mozione che dovevamo votare in Aula, quando ci siamo scontrati tra maggioranza e opposizione, oggi i toni sono cambiati. toni sono cambiati. Ci stiamo confrontando senza scontri e senza arrivare a contrapposizioni muro contro muro. Ognuno ha la sua tesi, la maggioranza è unita e sta portando avanti le sue idee all'interno di questo provvedimento

(*Segue* PORETTI). Si nega l'evidenza; si nega il codice deontologico. L'appello alla ragione non è stato colto dalla maggioranza, dal Governo e neppure dalla Presidenza del Senato, con quelle preclusioni che hanno falcidiato numerosi emendamenti. Purtroppo, non possiamo e non riteniamo neanche utile obbligarvi alla ragione: quest'obbligo di trattamento lo lasciamo alla maggioranza, che decide di obbligare

l'«io non lo farei» non può diventare il «tu non lo devi fare, e non lo devi fare per legge». Entrando nel merito dall'articolo 1

che si nega una legge sul testamento biologico: in quel primo comma si afferma infatti che la vita umana è indisponibile. Il diritto alla vita diventa l'obbligo di vita e alle condizioni che questa maggioranza e questo Senato stanno decidendo. Utilizzeremo poco tempo per illustrare gli emendamenti; ne prenderemo di più per svolgere delle dichiarazioni di voto a titolo personale, come singoli

rafforza il valore di indicazione costituzionale dell'elencazione contenuta nell'articolo 1.

scusi, senatore. Onorevoli colleghi, per cortesia, vi prego di abbassare il tono della voce nei dialoghi che state intrattenendo oppure di svolgerli all'esterno. Consentite al senatore

Per quanto riguarda l'emendamento 1.127, tutta la materia del consenso informato è già sufficientemente

non a tutta l'attività medica che, notoriamente, è ben più ampia e non sempre dipende da un consenso informato perché non sempre riguarda atti diagnostici e terapeutici sui pazienti. Ci sembrava opportuno in questa sede essere più precisi nell'indicare a quale consenso informato si facesse

rappresentano i criteri fondamentali a cui la legge deve ispirarsi. A tal proposito cito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, resa nel 2002 nel caso "Pretty -United Kingdom".

Passo più approfonditamente all'emendamento 1.206, su cui mi permetto di insistere fin da ora per il voto segreto. Questo emendamento mira a rendere la norma costituzionalmente legittima sotto il profilo del rispetto dei princìpi di tassatività, determinatezza e precisione della norma incriminatrice, espressi dall'articolo 25 della Costituzione.

L'emendamento 1.255 inserisce l'ulteriore richiamo alla tutela della dignità umana, nella parte dell'articolo 1 in cui si sancisce che la legge «garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati». II richiamo alla tutela della dignità e all'osservanza dei «limiti imposti dal rispetto della persona umana» (articolo 32, secondo periodo del secondo comma, della Costituzione) rappresenta infatti un parametro ermeneutico necessario per sancire espressamente l'illegittimità di ogni trattamento sanitario che, anche se privo dei requisiti di sproporzione o accanimento terapeutico già richiamati dalla norma, sia comunque incompatibile con la dignità umana. Tale precisazione è imprescindibile in quanto si presta a coprire tutta quell'area di trattamenti sanitari ancorché non configurino ipotesi di vero e proprio accanimento terapeutico, siano tuttavia lesivi di uno dei princìpi fondamentali - o meglio il metaprincipio fondativo della Costituzione, nel suo impianto personalistico quali la dignità umana. Si tratta di un riferimento tanto più importante ove si consideri che proprio il rispetto della dignità umana ha rappresentato uno dei motivi in base ai quali la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (ma anche la giurisprudenza di Strasburgo)

di una clausola riassuntiva che copre anche i diritti non scritti. Il diritto alla vita è un diritto non scritto della Costituzione. Per carità, il diritto c'è ed è riconosciuto e la Corte costituzionale lo ha inserito tra i diritti fondamentali; non si può prendere un diritto e dichiarare che a quello si deve sacrificare tutto, per di più quando si tratta di un diritto non scritto. Tutti i diritti inviolabili e i diritti fondamentali sopportano limitazioni, soprattutto quando possono andare in rotta di collisione due diritti fondamentali.

1.55. Si può anche sostenere che il diritto alla vita sia indisponibile anche per il soggetto, ma fino alla morte naturale, cioè fino al termine di un percorso chiaro ed identificato e non a una prosecuzione artificiale

il ragionamento di connessione con gli articoli del codice penale è molto pericoloso perché viola l'articolo 25 e crea un'indeterminatezza totale. L'emendamento 1.205

mira a recuperare il "soprattutto", che è scomparso, perché quel tipo di interventi che si proibisce nel caso di condizioni di morte prevista come imminente, se li definiamo non proporzionati o configurabili come accanimento terapeutico, vanno respinti "soprattutto" in quei casi, ma non solo.

al diritto inviolabile ed indisponibile della vita, anche "nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge", con il diritto "inviolabile e indisponibile

si "riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza".

individuali, le libertà inviolabili e soprattutto il diritto codificato nell'articolo 32 della Costituzione, per cui si può arrivare anche a rifiutare cure che possono salvarci la vita. Come preannunciato dalla senatrice Poretti, interverremo nuovamente durante

Signora Presidente, il principio per cui ho proposto questi emendamenti riguarda fondamentalmente la questione dell'indisponibilità.

strana e, per me, totalmente inaccettabile nei confronti della tradizione costituzionale italiana. Non è scritto in nessun articolo della Costituzione che la vita è un diritto inviolabile e, soprattutto, indisponibile. Ceccanti ha illustrato poc'anzi come il diritto alla vita sia una parte non scritta dell'articolo 2 e questo risolve già brillantemente a nostro favore

Costituzione parla di diritti inviolabili dell'uomo e tali diritti hanno una configurazione vasta che richiede una cultura necessaria per riuscire a capirne l'ampiezza. Da ciò però non si può desumere, come se fosse un'operazione algebrica, la conseguenza di una indisponibilità della vita. Trovo che sia proprio il concetto di indisponibilità a rappresentare un elemento potente e insidioso di falsificazione. E non solo tale concetto non è scritto nella Costituzione, ma ricordo di passaggio che la parola «vita» compare per la prima volta nella Carta costituzionale nell'articolo 38 laddove si parla del diritto del lavoratore a vedere salvaguardata la vita di fronte a problemi di incidenti sul lavoro. Quindi una via totalmente secondaria del ragionamento che non ha nulla a che vedere con il principio della vita come principio globale primario. Si

di una legge venga inserito un concetto pericolosissimo, ed ora spiego il perché. Se si sostiene che la vita è indisponibile per il soggetto che la vive vive rimane come sospeso - tra l'altro, in modo ipocrita, subdolo e non chiaro - il criterio che sarà disponibile per qualche autorità superiore, altrimenti non ci sarebbe bisogno di dirlo. E quale sarà mai questa autorità superiore? O Dio o lo Stato. In una legge non si può scrivere che la vita è indisponibile per l'uomo perché è disponibile per Dio: Dio: sarebbe un'intromissione indebita, il profilarsi di una dimensione di Stato teocratico. Il problema è che rimane solo lo Stato. Allora, la vita è disponibile solo per lo Stato. Dentro questo criterio per cui la vita non è disponibile per l'individuo che la vive, ma è disponibile invece per lo Stato si annida una ferita pericolosissima dal punto di vista del principio concettuale. Siamo di fronte al venir fuori di un'idea dello Stato etico di antica memoria, inteso come Stato coercitivo che impone al cittadino modi di pensare, obiettivi di vita, modi di relazione. un principio che considero pericolosissimo contro cui bisognerà battersi anche sul piano dell'opinione pubblica, se questa legge accetterà una simile formulazione. Tra l'altro è una formulazione inedita, non è mai esistita da nessuna parte. Sarei curioso di sapere chi l'ha inventata. Da dove viene fuori l'idea della vita indisponibile? Chi ha mai partorito questa stranezza? Dove l'hanno pescata? In quali testi l'hanno trovata? Non c'è da nessuna parte.

Per brevità, concordo con quanto detto poc'anzi dal senatore Pardi; aggiungo soltanto un'indicazione, e cioè che questa precisazione potrebbe essere surrettizia o addirittura subdola

sia indisponibile, o se soltanto per le persone diverse dal titolare; e allora si apre ancora la strada ad una volontà o ad una possibilità di punire eventualmente il tentato suicidio, con tutto quello che ne conseguirebbe.

proponiamo che venga indicato «di intendere o di volere», perché si tratta indubitabilmente di due categorie diverse di persone. Infatti, le scienze giuridiche e psichiatriche hanno ampiamente descritto che una qualità riguarda l'intelletto e l'altra riguarda la volontà e quindi credo vadano tutelate tutte le persone deboli, in quanto tali incapaci di intendere o di volere. Sull'emendamento 1.88 è già intervenuto il senatore Ceccanti, condivido l'impostazione: credo non abbia senso l'espressione «fino alla morte accertata nei modi di legge» e che si possa scrivere «fino alla morte naturale». Inserire l'espressione «nei modi di legge» crea sicuramente problemi interpretativi e darebbe adito a contestazioni, soprattutto davanti all'autorità giudiziaria.

la questione relativa alla eutanasia da quella che trattiamo con questo disegno di legge: sono due cose diverse e non vanno trattate in questo testo.

che il diritto alla vita umana vada garantito anche nella fase terminale dell'esistenza, perché questa dizione può far generare il sospetto, la presunzione che gli operatori sanitari non si comportino,

molto più chiaramente princìpi come quelli del consenso informato e un principio cardine come quello dell'autodeterminazione. Su due lettere vorrei accentrare maggiormente la vostra attenzione: la lettera *b)*, in cui si "riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza". Sinceramente non riesco a capire

la lettera *d)*, in cui sembra quasi che il paziente debba sforzarsi ad identificare consapevolmente le cure cui sottoporsi con la partecipazione del medico.

di fine vita; secondo noi il consenso informato è un principio dello stesso valore in tutte le fasi della vita. Quindi, col nostro emendamento 1.143, molto più semplice

scienza abbiamo parlato anche in Commissione riguardo ad un articolo per grandissima parte condiviso nella formulazione. Su questo vi erano state delle osservazioni, ritenendo che riferirsi alla scienza in generale potesse non coprire un campo di applicazione diretta sulla persona; ci siamo riferiti esattamente alle eventuali applicazioni che potessero essere usate sulla integrità stessa del soggetto e al di là della sua volontà. Quindi, ogni persona deve essere garantita totalmente nella sua dignità in modo prioritario, anche rispetto a qualsiasi interesse scientifico,

peculiare, soprattutto nel momento della fase di fine vita, vogliamo soltanto sottolineare che nel momento in cui vi potesse essere anche la incapacità del paziente a percepire in modo attivo questo rapporto, riteniamo che allora si esalta la lealtà di un rapporto fondamentale tra il medico ed il paziente.

si considerano e sono da tutti considerati come trattamenti inefficaci, inutili, spesso invasivi, a volte dannosi. Non capisco perché questi trattamenti, che vengono giustamente evitati nel caso delle persone in fin di vita, non dovrebbero essere evitati anche nei casi di un idraulico di 35 anni o di un bambino di 12 anni. Con l'emendamento

una particolare riflessione all'Aula sull'emendamento 1.251, che nonostante sia particolarmente sintetico credo debba meritare qualche riflessione. È un emendamento che punta ad una migliore definizione del concetto di accanimento terapeutico. Al di là della divisione che c'è in Aula tra chi tutela l'indisponibilità della vita e chi, al contrario, tutela il principio dell'autodeterminazione, tutto il provvedimento legislativo si concentra su due questioni molto semplici: la definizione dell'accanimento terapeutico e se esso comprenda o meno l'alimentazione e l'idratazione artificiale. Vorrei allora fare una considerazione sull'accanimento terapeutico, che fa comprendere la base dell'incostituzionalità di questa legge. legge. Noi definiamo l'accanimento terapeutico, signora Presidente, non per le persone che hanno capacità di intendere e di volere, non per le persone che hanno coscienza. anche se in questa legge viene scritto che l'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale, sin quando io ho piena coscienza e capacità di decidere e di intendere e di volere non ci potrà essere nessuna legge di Stato, nessun medico all'interno di una struttura sanitaria pubblica che mi potrà infilare per forza un sondino nasogastrico; lo dice la Costituzione e lo dice il codice deontologico. D'altra parte, l'onorevole Roccella sa che nel nostro Paese esistono 200.000 casi di pazienti affetti da anoressia mentale, patologia che colpisce soprattutto giovani e soprattutto donne e che ha un alto tasso di mortalità; cosa facciamo, sostenendo il principio che l'alimentazione e l'idratazione sono forme di sostegno vitale: sottoponiamo queste pazienti ad un trattamento sanitario obbligatorio e infiliamo loro un sondino nasogastrico?

L'accanimento terapeutico serve allora a chi non ha più capacità d'intendere e di volere. Ecco quindi già la base dell'incostituzionalità di questa legge, che fa una duplice distinzione tra i cittadini che hanno la capacità di decidere e che possono avere un trattamento diverso, nella legge, nella Costituzione e nei fatti, nel comportamento medico e di qualsiasi ospedale. Sono 25 anni che faccio il medico, ho girato ospedali di tutta Italia e non ho mai visto un paziente che non vuole alimentarsi e che viene bloccato da due infermieri, da un lato e dall'altro, con altri due infermieri che gli reggono le gambe, e che gli infilano un sondino nasogastrico.

Nonostante il relatore abbia detto questa mattina che la legge è chiara e semplice, con grande rispetto per chi vi ha lavorato e vi ha impiegato mesi e mesi di lavoro, io la considero ambigua e confusa. Qui definiamo l'accanimento terapeutico, prevedendo che il medico debba astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati. È una frase che dice tutto ed il contrario di tutto. È una frase di un'ambiguità che è in contrasto

sia nel 1995 che nel 2006, hadato una definizione ben precisa, prevedendo che il medico debba astenersi dall'accanimento terapeutico,

Questa è la definizione che l'Ordine dei medici ha dato dell'accanimento terapeutico nel 1995, ribadendola nel 2006.

particolarmente significativa la definizione che di accanimento terapeutico viene data nel disegno di legge n. 1323 dei senatori D'Alia e Fosson. di legge stabilisce: «Il medico deve astenersi dall'instaurare o proseguire trattamenti sanitari non proporzionati, futili o inutilmente invasivi e non efficaci rispetto alle condizioni cliniche del paziente e agli obiettivi di cura». I proponenti del disegno di legge poi aggiungono: «Egli non ha l'obbligo di contrastare e ritardare ad ogni costo l'esito finale della malattia, ma piuttosto, nel rispetto del migliore interesse del paziente, ha il compito di accompagnarlo ed assisterlo verso la sua fine naturale». Questa definizione Probabilmente da allora alcune posizioni sono mutate anche per la necessità di portare avanti delle giuste battaglie